Signora Presidente, onorevoli colleghi, il motivo per cui, dopo essere stato alla Camera sono qui oggi pomeriggio lo conoscete benissimo: è per rendervi informati nei dettagli del luttuoso evento che ha colpito ancora una volta le nostre Forze armate, i nostri militari che, in ossequio alla decisione dell'ONU, sono in Afghanistan; la morte di un tenente degli alpini, il ferimento di quattro militari è notizia che purtroppo ci ha raggiunto. E voglio subito

il più possibile veloce e dando la nostra solidarietà alle loro famiglie. Non è un'espressione formale, ma sentita e vera: è un fatto che colpisce il Paese con la stessa intensità tutte le volte che - purtroppo sono tante

IdV)*. Signora Presidente, onorevoli senatori, veniamo ai fatti: li ricostruisco secondo quanto mi dettano le

e costanza), si è mosso un dispositivo composto da una colonna di 12 mezzi italiani e uno della *Afghan National Army* che stava facendo rientro verso la base di Shindand, nella provincia di Herat. L'operazione di supporto sanitario era stata pianificata e condotta dal comando della *Task force center* su base del 5° Reggimento alpini, di stanza a Vipiteno, che attualmente è schierato proprio a Shindand, la cui area di responsabilità si estende per oltre 30.000 chilometri quadrati e comprende 14 distretti e circa 1.600 villaggi. Alcuni sono piccolissimi villaggi, altri più consistenti. Alle ore 12,45, orario di Herat (in Italia erano le 9,15 del mattino), a circa 4,5 chilometri a Sud-Ovest di Adraskan, un mezzo Lince - mezzo che ormai abbiamo imparato tutti a conoscere, sappiamo cos'è - e precisamente il secondo dei veicoli italiani della colonna, preceduto da un altro mezzo italiano e, prima di questo, dall'unico mezzo afgano della colonna colonna che, sia detto per completezza, comprendeva anche un'ambulanza, è stato coinvolto nell'esplosione di un ordigno artigianale ubicato sotto la sede stradale. Il nostro mezzo, il Lince, era dotato di un apparato disturbatore disturbatore (jammer), uno di quelli che servono a disinnescare il comando elettronico a distanza. L'esplosione provocava la distruzione del mezzo e causava il decesso di uno degli occupanti e il ferimento degli altri quattro

nei centri sanitari più attrezzati. Sul posto veniva immediatamente mandato un plotone della Forza veloce di reazione, la squadra specializzata del Genio per le eventuali azioni di recupero e per le indagini del caso. Il militare rimasto ucciso a seguito delle ferite riportate nel corso dell'attentato, come già sapete, è il tenente, oggi capitano, effettivo al 5° Reggimento alpini di Vipiteno, e residente a Occhiobello, in Provincia di Rovigo. in volo, rientrerà in Italia nella serata di oggi, intorno alle ore 21: non è stato possibile prima, come invece doveva essere secondo le previsioni, perché il maltempo ha impedito al nostro aereo di atterrare e poi di decollare in tempo verso Ciampino, dove, ripeto, arriverà questa sera. Nell'attentato sono rimasti feriti: il caporal maggiore scelto Giovanni Califano, che è ricoverato presso il «Role 2» spagnolo di Herat,

nonché un trauma addominale, con rottura della milza e frattura del calcagno bilaterale (ieri, è stato trasferito presso l'ospedale americano di Ramstein in Germania, dove è assistito anche dal nostro personale, oltre che dai suoi familiari, che abbiamo provveduto a trasferire lì); il caporal maggiore Salvatore Saputo, attualmente ricoverato presso l'ospedale da campo «Role 2» spagnolo di Herat, dopo essere stato ricoverato

inoltre sottoposto ad un piccolo intervento per estrarre un piccolo corpo estraneo da un occhio: anche per lui si sta organizzando l'evacuazione sanitaria in Italia); Italia); il caporale Mario Manfrin, ricoverato presso l'ospedale da campo «Role 2» di Herat, dopo essere stato ricoverato in quello statunitense di Shindand, ha riportato la frattura scomposta del femore destro, trattata chirurgicamente (è il militare che in un primo momento sembrava, o era, il più seriamente ferito dei quattro: anche per lui si sta organizzando la successiva evacuazione sanitaria in Italia). sono tutti effettivi al 5° Reggimento Alpini di Vipiteno e non versano fortunatamente in imminente pericolo di vita. Come appare evidente, le operazioni di soccorso sono risultate particolarmente complesse, sia per il numero di militari colpiti

in maniera encomiabile, l'evacuazione sanitaria, e mi riferisco non solo agli italiani, ma anche agli alleati, che hanno dato pieno sostegno, anche negli ospedali, ai nostri ragazzi feriti. Signora Presidente, onorevoli senatori, i fatti che vi ho descritto sono quelli che mi hanno riferito e che giungono dal teatro operativo.

devono aver fatto ricorso ad un ordigno diverso, ancora più antico se volete, tipo mina a pressione anticarro, o comandato via filo a distanza (ma tendiamo ad essere più orientati verso l'esplosione dell'ordigno a pressione, nel senso cioè che il peso del mezzo avrebbe fatto esplodere la forte carica). Come in tutti i casi simili, è stata disposta dal Capo di Stato maggiore della difesa un'inchiesta, e un'altra aperta dalla magistratura romana. Il Lince, ormai lo sappiamo - abbiamo imparato a conoscere questo mezzo - è un veicolo blindato concepito sulla base

lo chiamano scherzosamente San Lince. L'ultima occasione in cui ha prodotto un effetto positivo è stata proprio il 26 febbraio scorso, quando, nello stesso distretto di Shindand,

completamente distrutto la parte anteriore del Lince ma l'equipaggio non ha avuto danni (solo chi era in ralla si è fatto male ad un ginocchio, ma niente di serio). Anche a costo di allungare di qualche minuto la relazione, voglio darvi qualche nozione tecnica ulteriore. Nell'ambito delle misure tese al miglioramento della protezione e della sicurezza del personale, il Ministero, su indicazione del Parlamento (maggioranza e opposizioni) e con pieno accoglimento, lo voglio dire, del Ministro dell'economia e dell'intero Governo, ha sempre evidenziato con chiarezza l'esigenza che la sicurezza dei militari in missione di pace non venga commisurata alle esigenze di bilancio. Può essere commisurata alle esigenze di bilancio la misura della nostra proiezione, cioè il numero dei militari o la fattibilità della partecipazione ad una misura, non, una volta decisa la misura, le risorse necessarie a garantire il massimo della sicurezza.

la ricerca sulla sicurezza. Per esempio, dal luglio del 2010 sono stati immessi nel teatro afgano i primi 17 esemplari del veicolo blindato medio Freccia,

solo è di difficile manovrabilità, ma proprio non ci passa, o addirittura potrebbe sprofondare; ha però un uso complementare che è molto importante. importante. Aggiungo che, al fine di incrementare il livello di protezione del personale, sono stati acquisiti dagli Stati Uniti anche mezzi speciali, denominati Cougar, impiegati dai nuclei degli artificieri per il trasporto del personale e muniti della dotazione degli assetti,

sicurezza assoluta, in un teatro come questo. Ce lo insegna la storia: alla lancia si rispondeva con lo scudo, alle pallottole con la corazza, e via di questo passo. Naturalmente, più si intensifica la difesa e più chi chi vuole offendere è indotto ad aumentare la minaccia. Quindi non possiamo mai considerarci soddisfatti del livello di sicurezza raggiunto, ma bisogna continuare ad operare affinché vi sia sempre la disponibilità a dotare i nostri soldati di tutto ciò che è possibile,

di rischi. Signora Presidente, onorevoli colleghi, se questa è la parte relativa alla sicurezza, ciò che forse il Parlamento si aspetta

che, sono certo, almeno in questa occasione qualcuno chiederà. Quindi, dal punto di vista politico - strategico desidero in primo luogo ribadire con forza che in Afghanistan - spero di farlo per l'ultima volta in occasioni simili - la nostra presenza è finalizzata da sempre alla pacificazione e alla ricostruzione del Paese. Abbiamo fatto, a suo tempo, una scelta di campo tra democrazia e terrorismo. Ancora oggi rivendichiamo con orgoglio quella scelta e l'impegno in una missione internazionale nella quale, insieme agli alleati, agiamo per la sicurezza e l'assistenza del popolo afgano. La missione della NATO su mandato ONU - la nostra missione - non è quella di fare la guerra, ma non possiamo certo dividerci o fare polemiche su un termine lessicale o su una parola.

in tutti i modi, ma non credo che possiamo dividerci o impiccarci su una parola. L'articolo 11 della Costituzione - questo è invece importante - lo conosciamo benissimo. Me lo sono letto e riletto tante volte, dopo averlo studiato a scuola e all'università. Esso afferma che «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». È stato il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, a ricordarci che di certo l'Italia non è in Afghanistan per attentare alla libertà del popolo afgano. È stato il Presidente della Repubblica a ricordarci che l'Italia non è certo in Afghanistan per risolvere una controversia tra noi e lo Stato afgano. Semmai è vero esattamente il contrario:

avendo precise regole di ingaggio, collaborando con i Paesi alleati e avendo l'obbiettivo che tutti conoscono, quello di ridare al legittimo Governo afgano, in un regime di libertà e di democrazia, il controllo del territorio afgano.

un bombardamento a tappeto, un attacco preventivo di occupazione: cose che, a prescindere dalle finalità, sono esattamente l'opposto di come operano i nostri militari. Ricordo che, pur potendolo fare senza bisogno dell'autorizzazione di alcuno, per assicurare una maggiore condivisione del Parlamento ho anche disatteso una richiesta - per la verità non forte - della comunità della comunità internazionale, e quindi dei nostri militari, di dotare di bombe di precisione i nostri aerei. Ciò non significa, però, che non ci chiediamo ogni giorno come vadano le cose e cosa sia meglio fare. Anche il nostro Presidente del Consiglio, in dichiarazioni che sono state abbondantemente riportate, alla notizia della morte del tenente Ranzani ha detto che tutte le volte che succedono tragedie di questo tipo ci si chiede se questi sacrifici, che compiamo con il voto unanime del Parlamento e con il consenso degli italiani, siano sforzi che servono e che vanno in porto: egli ha detto che lo speriamo vivamente. La domanda che si pone il Presidente del Consiglio io me la pongo tutti i giorni. Ciascuno di voi se l'è posta più volte; a me tocca pormela di più, perché ogni giorno ho notizia di quello che succede, dei pericoli che corrono

abbiamo il dovere di dare una risposta, e non c'è domanda che non presupponga una risposta. La risposta che ci siamo dati e che ci diamo è semplice: la risposta è che siamo in quella missione per volontà del Parlamento italiano, in ossequio a una decisione internazionale, e che non abbiamo minimamente intenzione di assumere scelte unilaterali che costituiscano un *vulnus* del nostro rapporto con la comunità internazionale. È una decisione non difficile, perché non l'abbiamo mai neanche dovuta affrontare. Alla stessa domanda, rispondiamo che non lo facciamo solo per un vincolo

sarebbe la peggiore offesa non solo alla memoria di chi è caduto, ma anche al rispetto che dobbiamo a chi, anche in questo momento, mette in gioco la propria vita per adempiere al proprio dovere. E aggiungo: la risposta che diamo è conseguenza del convincimento che siamo lì non solo per dare libertà e democrazia al popolo afgano, alle donne, ai bambini e alle bambine ma anche per contrastare il terrorismo e per tenere il più lontano possibile dalle nostre case, dalle nostre città e dalle Nazioni della comunità internazionale il pericolo drammatico e concreto di un'espansione del terrorismo. È quindi una risposta dolorosa, che tiene conto naturalmente dei rischi, dei sacrifici, del dolore, della perdita di vite umane: certo che ne tiene conto! Tiene conto persino delle facili polemiche che possono derivare. Sarebbe comodo: c'è qualcuno che pensa che ci piaccia, che siamo contenti che ci sia questa situazione, e che non avremmo preferito che non ci fosse il pericolo del terrorismo, e quindi la necessità di questo intervento. Se c'è qualcuno che pensa Ma il dovere è quello di fare fronte alle emergenze esistenti. E poi ci chiediamo tutte le volte se queste vittime potessero essere, in qualche modo, evitate. E lì più difficile è la risposta, caso per caso. Certo è che è aumentato il rischio ed è aumentata la frequenza degli episodi di attacco. Ma tutti i dati in mio possesso questo dato estremamente doloroso è, non solo prevedibile, ma addirittura inevitabile, perché l'aumento del numero dei militari, la presenza massiccia sul territorio, la strategia, che abbiamo applicato, di cercare di far stare il più vicino possibile la fase della ricostruzione a quella del contrasto con la forza giusta dell'*insurgence* del terrorismo porta a un aumento della D'altronde, senza questa strategia sarebbe infinito il tempo che ci separa dal momento in cui potremo riconsegnare al legittimo Governo afgano, ai singoli governatori dei distretti, il territorio afgano. Non dovremo aspettare che sia venuta meno ogni minaccia, ma dobbiamo accelerare al massimo il momento in cui le minacce di questo genere potranno essere autonomamente contrastate dalle Forze armate afgane, dalla polizia afgana e la situazione potrà essere autonomamente gestita dal Governo afgano. A questo noi miriamo, e questo comporta un aumento di pericolosità, che non riguarda l'Italia: anzi, devo dire che, complessivamente, in questi anni il buon Dio (semmai una contabilità del genere avesse un senso) ci ha posto nella condizione di avere lutti enormi, ma quantitativamente inferiori a quelli, anche in proporzione, di altri Paesi. Ma non è certo questa una consolazione, né una contabilità che possa avere un senso. È giusto evidenziare anche - e me lo chiedeva un parlamentare i passi avanti concreti, dal punto di vista della ricostruzione che sta compiendo la missione. Non tanto i passi avanti in termini militari: noi parliamo, giustamente, solo dei lutti e diamo, volutamente, scarso rilievo ai successi di uso anche della forza giusta, della capacità di respingere 99 attacchi su 100. È ovvio che sia così, è normale: ma è giusto evidenziare almeno i successi nell'opera di ricostruzione. nell'opera di ricostruzione. Voglio farvi un piccolo esempio: solo uno, ma ce ne sono 100. Proprio lunedì scorso è stata inaugurata una scuola nel villaggio di Shakinban, nel distretto di Zindajan, sempre nella provincia di Herat, in vista del nuovo anno scolastico e grazie all'azione congiunta del PRT, cioè del *team* di ricostruzione gestito dall'Italia e dalla cooperazione italiana.

a studiare 1.383 alunni di età compresa tra i 13 e i 20 anni, per ottenere un diploma di istruzione superiore. Certo, è un piccolo segnale, ma è giusto comprendere che, senza l'uso della forza giusta, questi segnali non ci sarebbero, e neanche sarebbe più vicino il momento di riconsegna agli afgani. Ho riferito alla Camera, e voglio ripeterlo anche qui, che continuo ad insistere (ed abbiamo ottenuto risultati in tal senso) affinché la commissione che ha il compito di decidere quando ogni singolo distretto passerà agli afgani

C'è bisogno, e ci stiamo riuscendo, che si stabilisca che, quando la minaccia arriva a questi livelli, in quel momento scatta automaticamente la possibilità di riconsegna. Ripeto, infatti, che non ci aspettiamo certo

Voglio infine ricordare a tutti noi che parliamo in questa Aula del problema generale,

vi dia, in maniera assolutamente sincera, contezza dell'orgoglio, insieme alla solidarietà che provo per famiglie come quella del militare Miotto, scomparso poco tempo fa - ho ricevuto proprio ieri una lettera bellissima dalla madre che provo per la famiglia del tenente Ranzani e per lui stesso. Pensate a questo giovane che da ragazzo faceva il *boyscout*

merita non solo il nostro commosso ricordo, ma la nostra ammirata partecipazione alla sua scelta di vita. Ho concluso il mio intervento, ma desidero aggiungere una postilla come ho fatto alla Camera.

Grazie, Presidente. purtroppo ci troviamo sempre più spesso a dover subire, trattandosi di una ricezione di nozioni tecniche miste a notizie luttuose, informazioni relativamente alla presenza degli italiani all'estero nelle missioni di pace. Oggi abbiamo ancora una volta avuto molte nozioni tecniche con una conclusione da comizio, ma non c'è stata detta una parola, che fosse una, relativamente al contesto geopolitico e strategico dove sono avvenuti i fatti al centro dell'informativa. L'estate scorsa la 3a e la 4a Commissione del Senato all'unanimità avevano deliberato l'avvio di una indagine conoscitiva relativamente alla presenza italiana in Afghanistan; ebbene, sono passati otto mesi e non si è fatto un passo in avanti

Il Parlamento non è né un luogo dove si fanno conferenze stampa, né tantomeno un pensatoio da scuola di guerra, ma è un luogo dove si dovrebbe dibattere. Abbiamo adottato un ordine del giorno a stragrande maggioranza - anzi credo all'unanimità quando abbiamo rinnovato il mandato alle nostre missioni e il loro finanziamento in cui si chiede un quadro normativo preciso all'interno del quale dibattere nel merito le questioni relative all'opportunità e alla necessità di essere presenti nel mondo, non per riconsegnare agli afghani l'Afghanistan, ma per promuovere diritti umani, pace e democrazia, e quindi sicurezza internazionale. Se anche il Presidente del Consiglio, ogni volta che muore qualcuno, si pone il dubbio sulla nostra necessità di essere colà, credo che anche il Parlamento debba essere messo in grado di poterne dibattere approfonditamente.

bisogna solamente fare un apprezzamento e cercare di non mettere in discussione le situazioni. Non bisogna mai dividere una linea operativa, anche con la comunità internazionale: il Ministro ha sempre detto che ci sarebbero state recrudescenze durante l'anno, e sapevamo benissimo a che cosa saremmo andati incontro. Quindi, in questi momenti bisogna essere forti, anche in quelli di più grande dolore, visto che conoscevo personalmente il caduto. Il popolo italiano è un grande popolo ancora, fuori, e contribuisce alla pace e alla stabilità nel mondo con grande spirito di sacrificio, nell'interesse dei popoli in difficoltà.

intendo esprimere il dolore, mio personale e dei colleghi del Gruppo dell'Italia dei Valori, per la morte del tenente Massimo Ranzani. Vorrei anche rappresentare la vicinanza ai congiunti del tenente caduto, così come ai suoi colleghi che sono rimasti feriti insieme a lui.

ci ha detto che in questi momenti bisogna riflettere. Noi allora dobbiamo riflettere sul perché questi ragazzi muoiono. So che non condividerà il mio pensiero, che è quello del Gruppo e del Partito dell'Italia dei Valori; spero non chieda al Presidente di cacciarmi se non la penso come lei, e considero il suo discorso pieno di retorica. In questo Paese, signor Ministro, esiste la libertà di pensiero e di critica, non so se ne sia accorto. Le ricordo che l'Italia dei Valori chiede il ritiro delle nostre truppe non in occasione - come ha detto lei - di tragedie come queste, ma da quando non è più una missione di pace, da quando non è più diventata una missione di pace. Lei ha ragionato pronunciando una frase che ci fa preoccupare ancora di più: «Restiamo per i caduti».

giusto spiegarglielo, visto che lei ci tiene molto a precisare, come per l'articolo 11. Il termine «retorica», signor Ministro, indica un linguaggio ampolloso, ricco di orpelli ma povero di contenuti; e povero di contenuti è stato il suo discorso, perché non ha ricordato quello che poche ore fa il Presidente Karzai, con una secca frase, ci ha mandato a dire: la NATO e l'ISAF «devono concentrarsi sulle basi terroristiche e non sull'uccisione quotidiana di civili innocenti» (nove bambini tra i sette e i nove anni). Ragioniamo anche su questo, visto che

Peccato che da un mese a questa parte non abbia più le rassicurazioni neanche del suo Presidente del Consiglio, visto che ieri o l'altro ieri ha fatto, con nostra soddisfazione, un discorso quasi filo-dipietrista, dicendo che è ora di chiudere questo capitolo. Signor Ministro, lei dice che il venire meno, oggi, al nostro impegno sarebbe un tradimento per i nostri soldati. Noi dell'Italia dei Valori le ripetiamo che non è così. Ministro, lei lo sa bene che la posizione dell'Italia dei Valori è sempre stata chiara: abbiamo ribadito più e più volte il nostro convinto no alla permanenza delle truppe in Afghanistan.

Peccato che, nonostante l'inizio del 2011, siano in continuo aumento i militari che raggiungono l'Afghanistan (ben 4.200), e purtroppo sono in continuo aumento anche i caduti (già tre dall'inizio dell'anno). È per questo, signor Ministro, che le chiedo: quanti soldati dobbiamo ancora inviare per realizzare questa nostra *exit strategy*? Quante bare dobbiamo ancora accogliere a Ciampino con gli onori? Signor Ministro, noi vorremmo che si rimettesse in discussione la nostra partecipazione, perché gli sviluppi della stessa non sono più compatibili con il dettato della nostra Costituzione. Le ricordo l'articolo 11, che lei ha tenuto a leggere: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». Questo è il dettato dell'articolo 11, della mia e credo anche della sua Costituzione. Con 25 dei 35 morti caduti in azioni di combattimento, secondo voi in che situazione siamo oggi in Afghanistan? anche in conseguenza dell'articolo della Costituzione appena citato, ricordo che lei in questo Governo è il Ministro della difesa e, purtroppo per lei, non è il Ministro della guerra. Si adoperi, la prego, in modo da poter restare tale.

ringrazio il Governo per la puntuale e dettagliata descrizione dei fatti e mi associo, anche a nome degli altri componenti del Gruppo, al cordoglio per la morte del tenente, ora capitano degli alpini Massimo Ranzani.

è possibile fare una sintesi, cogliendo anzitutto la circostanza che è morto un soldato, un italiano che stava compiendo il proprio dovere. Non c'è quindi ripetitività inutile, né nelle comunicazioni del Ministro né in questo nostro intervenire. C'è, piuttosto, consapevolezza che ciascuno di questi morti restituitici dal difficile ambiente afgano rappresenta noi tutti, rappresenta l'Italia, che ha assunto un obbligo internazionale, secondo una prospettiva di pacificazione di un'area delicatissima, e lo assolve con dedizione totale. Per questo sono apparse improvvide le parole del Presidente del Consiglio che, commentando piuttosto superficialmente quest'ultimo luttuoso evento, ci ha voluto far sapere che ogni volta che accade qualcosa di simile si interroga se valga la pena essere là con nostri soldati. le scelte di politica estera sono uno dei pilastri di sostegno di un Governo democratico, e normalmente vengono dettate dal Parlamento con una certa solennità. Il Governo ne è promotore ed artefice, e può ovviamente orientare diversamente l'indirizzo del Paese in politica estera, ma, per quel necessario radicamento parlamentare, non può esimersi dal venire qui ad illustrare i motivi di un eventuale cambiamento. Sull'intervento in Afghanistan, non più tardi della settimana scorsa questo Senato ha convertito in legge il decreto-legge che ne prorogava il finanziamento, assieme alle altre missioni internazionali, sino al prossimo 30 giugno. È cambiato qualcosa? Se sì, è grave compito del Presidente del Consiglio informare il Parlamento e chiedere uno specifico appoggio; se no, come appare probabile ed utile, eviti il Presidente del Consiglio il facile ammiccamento al pensiero debole, nel quale purtroppo eccelle. Ne va del rispetto al dolore di una famiglia; ne va del rispetto al sentimento patriottico per il nostro caduto; ne va del rispetto alla qualità dell'impegno italiano sul fronte afgano e su tutti gli altri scenari ove sono dispiegati i nostri soldati; ne va della credibilità nazionale, già così compromessa su taluni versanti nell'opinione di molte Cancellerie del mondo. Sono le stesse Cancellerie presso le quali l'Italia si è invece consapevolmente accreditata per un intervento che coinvolge quasi 40 Stati, orientato a definire condizioni di sicurezza in un Paese nel quale possano così emergere percorsi di democrazia e di sviluppo. Le nostre truppe sono in Afganistan per aumentare le capacità operative dell'esercito e della polizia locali; per garantire sicurezza a quelle popolazioni; per ridurre le condizioni di incubazione del terrorismo internazionale. La grande coalizione alleata di sicuro non lavora perché questo complesso intervento duri indefinitamente. Non è questo, mi pare, il momento di scelte unilaterali che ci distinguano dai Paesi europei e dagli Stati Uniti d'America, a fianco dei quali siamo così significativamente impegnati. Noto che è la stessa conclusione dell'onorevole Ministro. Auspico linearità a venire e coinvolgimento immediato del Parlamento, ove le preoccupazioni comunque oggi emerse nell'intervento del Ministro dovessero modificare l'indirizzo governativo. Signora Presidente, signor Ministro, poche parole per esprimere a nome del mio Gruppo parlamentare il cordoglio per la morte dell'ufficiale degli alpini Massimo Ranzani; per esprimere solidarietà e vicinanza alla sua famiglia; per esprimere un affettuoso saluto ai quattro militari feriti, con l'augurio di una pronta guarigione; per ribadire, senza alcun tentennamento, il nostro sostegno a questa e alle altre missioni internazionali umanitarie e di pace; per ribadire il nostro ringraziamento ai militari che operano in quell'area con grandi difficoltà, tali per cui, come è stato ricordato, il Parlamento ha aumentato anche lo stanziamento finanziario relativo alla missione. È oltremodo evidente che noi da quell'area non possiamo andare via. A tutti piacerebbe indulgere a dichiarazioni come quelle che dicono che il nostro cuore vorrebbe portarci da un'altra parte, ma dobbiamo stare lì. Il nostro cuore e la nostra testa ci portano esattamente allo stesso posto, perché quando si ha cultura di governo e ci si assume la responsabilità di alcune scelte, queste devono essere portate fino in fondo, senza presunti sdoppiamenti di personalità che non fanno bene al Paese e che non danno peraltro una buona immagine anche di

fastidio e non fossero utili in Afghanistan, e se la gente afgana non si fidasse di noi, è evidente che nessuno ci presterebbe certe tragiche attenzioni. Se i talebani, i terroristi, ci fanno oggetto di attentati, significa che la nostra presenza lì produce effetti positivi ai fini della stabilizzazione del Paese e del suo ritorno alla normalità e alla democrazia. Se così è, credo che il Parlamento abbia il diritto e il dovere di conoscere fino in fondo

Presidente, signor Ministro, innanzitutto mi vorrei scusare

Secondo noi non sono questi i momenti per fare polemiche. Può anche essere vero che altre persone sono morte per la pace, ma non è togliendo dignità a chi è morto con un'arma in mano che si estende dignità ad altre persone che per lo stesso fine hanno dato la vita. Va detto poi che i nostri militari sono là non per fare la guerra, ma per ricostruire - questo è l'obbligo del contingente italiano

Il nostro obiettivo è infatti esportare e far conoscere la democrazia e le libertà, aspetti che sembrano scontati ma che lo sono solo per noi occidentali.

quel Nord Africa ormai in fermento, prendessero piede i partiti fondamentalisti islamici. Probabilmente non sarebbe più tutto come prima,

Lì in Afghanistan i nostri militari danno anche la loro vita, ma lo fanno per far sì che le nostre libertà e le nostre conquiste non siano domani poste a rischio: caro collega Pedica, non sono lì per altri motivi. Ogni tanto qualcuno lo piangiamo anche, ma lo facciamo per non dover piangere molte centinaia - e in America migliaia - di vittime in casa.

Appena qualche giorno fa noi abbiamo votato a favore del provvedimento di proroga delle missioni internazionali: lo abbiamo fatto con convinzione, pur essendo portatori di dubbi e perplessità, che però abbiamo ritenuto di dover espungere al momento della votazione, in ragione del fatto che rispetto a questo argomento ci si deve porre e disporre con estrema serietà. Questa serietà può essere chiamata anche sobrietà, signor Ministro, e io mi permetto sommessamente di invitarla a questa sobrietà, perché quanto ha riferito stasera avrebbe potuto dirlo anche senza incorrere in un tono enfatico e retorico, del quale francamente non c'è bisogno. Non c'è la necessità

richiamato, signor Ministro, noi abbiamo ribadito che quel voto era strettamente collegato al rispetto del mandato del Parlamento. Su questo argomento, signor Ministro, sono tre anni che la invitiamo a venire in quest'Aula per discutere con noi, e io sono lieto di averla sentita ripetere per l'ennesima volta che il rapporto tra il Governo italiano e la comunità internazionale, ma anche fra il Governo italiano e il suo Parlamento (o meglio il Parlamento del popolo italiano) non deve svilupparsi soltanto in occasione di queste tristi vicende: in buona sostanza, questa non in buona sostanza, questa non deve essere una sorta di orazione funebre ammantata di una spolveratina di ragionamento politico. Ed è per queste ragioni che noi le rinnoviamo l'invito: si venga in Parlamento e si ragioni non occasionalmente. Lei stesso, signor Ministro, ha detto appena pochi minuti fa che preferirebbe evitare che in queste circostanze si ragionasse di politica internazionale. Noi accediamo al suo invito, evitiamo in questa sede di parlarne, ma le chiediamo di impegnarsi perché questa benedetta dichiarazione di disponibilità si trasformi in un atto concreto. Venga nel mese di marzo corrente (quindi 2011) in Parlamento per ragionare con noi rispetto alla sua attività diplomatica con gli altri Paesi coinvolti nelle missioni internazionali

la nostra non scontata ma sentita ammirazione, pur senza sentire il bisogno di perderci in atteggiamenti di pedissequa accettazione di cose peraltro non richieste, come abbiamo avuto modo di verificare recentemente prendendo conoscenza di certi atteggiamenti tenuti dal Presidente del Consiglio, sia in occasione

*(PD)*. Se non mi guarda, vuol dire che non mi sta ascoltando.

la sollecitudine che l'urgenza impone, sollecitare appunto il presidente Schifani affinché possa adeguatamente rappresentare

sull'andamento della missione internazionale in Afghanistan. Questo, per essere chiari, non comporta minimamente la messa in discussione delle nostre scelte. Noi abbiamo votato con convinzione, e la convinzione la confermiamo. Chiediamo però che il Governo non incassi il nostro voto tutte le volte come qualcosa di scontato, del quale dimenticarsi il giorno dopo per ricordarsene dopo sei mesi alla vigilia della votazione del nuovo provvedimento. Le missioni internazionali, signora Presidente, non sono un fatto di ragioneria,

Signora Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il ministro La Russa, la cui disponibilità al confronto con il Parlamento è nota, per l'approfondita ed esaustiva relazione sui fatti che il 28 febbraio hanno portato alla morte del tenente degli alpini, Massimo Ranzani, alla cui famiglia va l'affettuoso cordoglio e la commossa solidarietà di noi tutti. Ma ringrazio il Ministro anche per aver voluto ribadire il senso della nostra missione in Afghanistan. Vedete, è in momenti come questi, segnati dal dolore e attraversati da inevitabili inquietudini, che abbiamo l'obbligo di essere fermi, coerenti e rigorosi o, per dirla altrimenti, che abbiamo l'obbligo di essere seri. So bene che il tenente Ranzani è la trentasettesima vittima italiana in terra afgana dall'inizio dell'intervento militare a fini di pace, e so che il suo nome, andando ad aggiungersi a quelli degli altri compatrioti lì caduti, compone oggi un tragico rosario che la nostra memoria sgrana con crescente angoscia. anche che, quando un soldato muore adempiendo al proprio dovere, alla politica spetta soprattutto il compito di onorare quel sacrificio, riaffermando tutte quelle ragioni che non lo rendono vano: ragioni che il ministro La Russa ci ha nuovamente illustrato oggi. Non si tratta, colleghi, di tacitare gli eventuali dubbi o i legittimi interrogativi della politica con un ricorso alla retorica, come sostiene, erroneamente e superficialmente, qualcuno: non Si tratta, piuttosto, di dare alla politica consapevolezza della propria responsabilità, perché questo, anche per la politica, è il tempo del dovere, il dovere di essere vicini alle nostre Forze armate e di essere uniti come italiani, per continuare a sostenere - come ha fatto finora positivamente il Parlamento - il processo di stabilizzazione e di democratizzazione dell'Afghanistan, in accordo con la comunità internazionale e nel rispetto degli impegni assunti con la NATO e con le Nazioni Unite. Poi verrà pure per la politica, senatore Scanu, il tempo del diritto alla riflessione, del diritto all'analisi e alla valutazione delle modalità e dei risultati delle missioni internazionali, specie alla luce dei profondi mutamenti geopolitici che si stanno verificando nell'area del Mediterraneo, la cui portata non potrà non incidere sulle priorità strategiche del nostro Paese e dell'Alleanza atlantica. lo ripeto, ci troviamo a vivere soprattutto il tempo del dovere, ed è allora nostro precipuo dovere dar prova di determinazione e coesione nazionale nel contrasto al terrorismo internazionale, onde ridurre la pressione dei talebani sui nostri soldati. noto, infatti, che in Afghanistan alcuni gruppi di insorgenti cercano di bersagliare sempre più i contingenti di quelle Nazioni da loro considerate maggiormente vulnerabili ai cedimenti del consenso interno, nell'intento di ottenerne il ritiro. Un calcolo che, per quanto ci concerne, si è fortunatamente rivelato sbagliato, perlomeno finora, visto che l'Italia non solo partecipa convintamente alla missione di stabilizzazione economica, sociale ed umanitaria in Afghanistan, ha anche recentemente prorogato e rifinanziato la partecipazione delle sue Forze armate e di polizia alle missioni internazionali sotto l'egida dell'ONU. vorrei ricordarlo - servono a perseguire obiettivi di pace e di libertà e a rinsaldare, sia pure in una logica multilaterale, i vincoli del nostro sistema di alleanze, facendo di questo stesso sistema, così rafforzato, un oggettivo moltiplicatore dell'influenza e del prestigio italiani, il che ci consente di sedere autorevolmente a tavoli politici ove poter ottenere vantaggi in termini di sicurezza e di geoeconomia. Capisco perciò, colleghi, i moti del cuore che esaltano il genuino sentimento di umanità ferita dinanzi al sangue versato, ma credo che questa nobile sensibilità debba essere tenuta a freno, dalla ragion politica prima ancora che dalla ragione di Stato, per quel senso di responsabilità che deve portare il Parlamento a privilegiare l'interesse generale della sicurezza dell'Italia. Esprimere quindi il nostro cordoglio con il linguaggio della ragione e fare il nostro dovere, rispettando le storiche alleanze e mantenendo fede agli impegni presi in sede internazionale, è allora il modo migliore per rendere onore alla memoria e al sacrificio del tenente Ranzani. La Patria gli sia grata.

Onorevoli colleghi, Onorevoli colleghi, con lettera in data 1° marzo 2011, pervenuta in data odierna, i senatori Cardiello, Carrara, Castiglione, Menardi, Palmizio, Piscitelli, Poli Bortone,

vice capogruppo il senatore Villari e tesoriere il senatore Piscitelli. Conseguentemente, Conseguentemente, i senatori Cardiello, Carrara, Palmizio e Piscitelli cessano di appartenere al Gruppo del Popolo della Libertà; Libertà; i senatori Menardi, Saia e Viespoli cessano di appartenere al Gruppo Futuro e Libertà per l'Italia; i senatori Castiglione e Villari cessano di appartenere al Gruppo Misto;

il Gruppo Futuro e Libertà per l'Italia è dichiarato sciolto, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del Regolamento. Entro tre giorni da oggi, i restanti componenti del Gruppo hanno facoltà di aderire ad altri Gruppi; decorso tale termine, saranno iscritti al Gruppo Misto.

così importante quale quello dell'educazione in relazione al problema del prezzo dei libri. vorrei fare solo una precisazione di carattere burocratico. Lei ha comunicato i nomi dei membri del Gruppo Futuro e Libertà che hanno aderito al nuovo Gruppo e ha fatto riferimento alla circostanza che in tre giorni gli altri hanno la possibilità di fare un'opzione. Per precisione, vorrei specificare che il senatore Pontone ha già presentato la sua opzione, che è stata comunicata all'Aula, nei confronti del Gruppo del Popolo della Libertà.

«La 1a Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione per il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

Questo disegno di legge decide di promuovere i libri mettendo dei paletti alla possibilità di fare degli sconti,

a favore della liberalizzazione degli sconti, e quindi anche della possibilità della liberalizzazione del prezzo dei libri,

concludo questo mio intervento con un piccolo racconto, che abbiamo ripreso da un *focus* dell'istituto «Bruno Leoni».

dove c'è questa liberalizzazione selvaggia, è iniziata una vera propria guerra tra i vari rivenditori; il prezzo, da 18 sterline, è crollato a 5 sterline. Una vera e propria guerra al ribasso. È successo che anche le piccole librerie e i piccoli rivenditori hanno preferito azzerare il margine di guadagno, o addirittura vendere sottocosto,

che noi vogliamo tutelare con il prezzo fisso e con lo sconto fisso, in realtà nella perfida Inghilterra, dove gli sconti sono liberi, sono sopravvissute con queste modalità. Si potrebbe dire: giù il prezzo e su le vendite. Vi invitiamo pertanto a votare i nostri emendamenti. Mi auguro che questo provvedimento, anche anche se *bipartisan*, venga guardato con un occhio di riguardo. Non è detto che intervenire così pesantemente sul mercato poi alla fine tuteli il consumatore, l'utente, colui che va a comprare il libro. Sicuramente così si tutelano anche le grandi distribuzioni e

che siamo dentro un sistema di equilibrio complesso tra un intervento regolatorio e il mercato: dico questo anche per fornire un'implicita risposta alla pur brillante esposizione della collega Poretti. Non c'è un inno allo statalismo e non c'è un inno al liberismo: si tratta di un tentativo regolatorio di buonsenso, in chiave europea.

«Al fine di valutare gli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, decorsi dodici mesi dalla loro entrata in vigore, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dei beni culturali, nel quadro delle rispettive competenze, trasmette una relazione alle Camere sugli effetti delle predette disposizioni sul settore del libro».

dalle posizioni politiche stesse o addirittura ideologiche. La conferma è che anche oggi il nostro Gruppo vota compatto a favore di tale provvedimento. La proposta di legge, già approvata in sede deliberante dai colleghi della Camera dei deputati, intende disciplinare le modalità con le quali si determina il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale e i limiti agli sconti che possono essere praticati rispetto al prezzo già determinato. Ad oggi, la disciplina vigente è dettata come è noto a tutti - dall'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, riguardante le norme sull'editoria e sui prodotti editoriali, che ha modificato anche la legge 5 agosto 1981, n. 416. Ci pare opportuno ricordare ancora che, di fatto, il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare rappresenta una piccola parte, un articolo di quello che era il progetto di rivisitazione della materia "editoria" che lo scorso Governo si era preoccupato di approntare, ma che non poté portare a compimento a causa della fine anticipata della legislatura. E non è certo un caso che su tale provvedimento si sia registrata anche la convergenza degli editori e dei librai, i quali ritengono il medesimo un compromesso tra le rispettive posizioni a riguardo dei modi attraverso cui arrivare alla determinazione del prezzo dei libri. Attualmente si opta per una via di mezzo tra i due modelli esistenti - l'uno prevede l'impossibilità di praticare sconti; l'altro prevede di fissare liberamente il prezzo di vendita dei libri sul mercato - attuando politiche di promozione sul prezzo e sconti applicati, ma senza che viga una disciplina certa a riguardo. L'obiettivo che si è prefisso di raggiungere questo disegno di legge è di far individuare liberamente il prezzo di vendita agli editori, prevedendo quindi dei periodi promozionali realizzabili durante l'anno solare - ai quali i librai potranno non aderire - e infine stabilendo un tetto massimo alla scontistica applicabile. All'articolo 1 della presente proposta di legge si sanciscono con chiarezza l'oggetto e le finalità generali dell'intervento legislativo. All'articolo 2, comma 1, si attribuisce all'editore o all'importatore il diritto di stabilire il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale. Il comma 2 prevede il limite massimo al quale attenersi per applicare la scontistica sul prezzo di vendita al consumatore finale, indipendentemente dalle modalità di vendita. Il comma 3 riconduce al potere di determinazione del prezzo di vendita da parte dell'editore o dell'importatore anche la possibilità di realizzare campagne promozionali che prevedano sconti a vantaggio del consumatore finale, salva la facoltà del rivenditore al dettaglio di non aderire a tali campagne. Nei commi successivi è stato quindi disposto circa il tetto massimo applicabile in determinate situazioni, quali manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, regionale, locale o se in favore di associazioni non lucrative, o ancora in altri casi specifici individuati dal legislatore. Su queste variabili la Commissione ha approvato delle modificazioni rispetto al testo licenziato dalla Camera e su queste erano concentrati gli emendamenti presentati per la discussione del provvedimento. Il Gruppo dell'Italia dei Valori è favorevole alla procedura per stabilizzare i prezzi dei libri individuata con questo provvedimento ed è per questo che annuncio il nostro voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo

il testo che ci accingiamo ad approvare offre un punto di equilibrio e di sintesi tra le diverse esigenze di un mondo, come quello del libro, popolato da attori tra loro estremamente diversi per interessi, per dimensione, per capacità e potenza finanziaria, fatto da librai ed editori. Il provvedimento, quindi, quale punto di sintesi tra istanze molteplici, pur essendo un importante punto di arrivo, deve contestualmente rappresentare anche un punto di partenza per avviare un lavoro che dovrà iniziare sin da subito, al fine di disciplinare una più vasta regolazione del settore attraverso quella legge generale sul libro che già esiste in altri Paesi e di cui l'Italia avrebbe tanto bisogno per promuovere la lettura attraverso scuole e biblioteche.

Nonostante si rilevi un vasto consenso sul provvedimento, bisogna tenere in conto che il mondo delle librerie, dei librai e delle case editrici è molto diversificato e differenziato tra grandi, medi e piccoli, con realtà regionali diverse, con situazioni differenziate che vanno tenute in considerazione. Questa variegata realtà si riflette anche sull'aspetto promozionale e sulle campagne a favore dell'impulso alla fruizione del libro e della lettura. Troppo spesso, infatti, se ne sono avvantaggiati i grandi e poco si è fatto per l'impulso della piccola editoria o dei giovani autori. Per quanto riguarda il metodo, formulo il mio apprezzamento e quello del mio Gruppo per il lavoro fatto in Commissione per giungere in modo concorde a un'intesa. Credo inoltre che l'ampia consultazione, che è stata effettuata propedeuticamente alla formulazione di questo testo, non solo ha permesso di arrivare all'elaborazione di una proposta condivisa, ma ha anche consentito di confermare l'idea di quanto sia importante, in società articolate, mettere in atto strumenti di partecipazione ampia e diffusa. Le recenti prese di coscienza e i conseguenti movimenti di rivolta a regimi dittatoriali nel Nord Africa sono dovuti anche all'accesso delle nuove generazioni ai mezzi di informazione e alla cultura in genere. Nel nostro Paese l'editoria è la prima azienda culturale nazionale, di gran lunga più forte e più diffusa del cinema, del teatro, dell'*home video*. Abbiamo un ricavo annuo di oltre 3 miliardi. Non siamo ai livelli di Germania, Francia e Regno Unito, ma ci annoveriamo fra gli otto mercati più forti al mondo. La distanza che ci divide dagli Stati Uniti, dal Giappone, dalla Francia, dalla Germania e dal Regno Unito tuttavia è ampia. Ciò ci deve indurre ad una legislazione più incisiva a sostegno dell'editoria, delle librerie, dei piccoli e medi editori. Questa legge si propone di aiutare il settore. Si è partiti da una ricognizione molto precisa delle esperienze europee, da quella tedesca a quella del Regno Unito, modelli abbastanza diversi per individuare possibili soluzioni in un modello intermedio, simile a quello francese. Si è deciso di regolamentare le campagne promozionali che sono certamente positive, ma dovevano essere disciplinate, e si è fissato uno sconto possibile che vada incontro alle esigenze sia degli editori che dei clienti. L'obiettivo è quindi quello di riordinare un settore laddove la confusione regnava sovrana. Sia sul merito che sul metodo, quindi, mi sento di poter dire che è stato fatto, tutti insieme, un buon lavoro. Incrementare la lettura e la possibilità che tanti cittadini italiani leggano è oggi più che mai fondamentale per la crescita culturale e civile del nostro Paese, e non solo. Credo inoltre che questa legge sia importante proprio perché di iniziativa parlamentare (visto che ne abbiamo tanto poche), e perché, pur non prevedendo maggiori oneri a carico della finanza pubblica, concorre a risolvere una questione importante del Paese ovvero introduce elementi di promozione di un settore attualmente in sofferenza. Nel dichiarare pertanto il voto favorevole del mio Gruppo a questo provvedimento, auspico un'approvazione corale e un impegno unitario per una legge di sistema che possa davvero dare un forte sviluppo complessivo al settore librario e, conseguentemente, anche alla creatività letteraria (soprattutto dei giovani) ed alla promozione del libro, che io ritengo, ma credo di interpretare un pensiero comune, possieda un forte spazio di attrattività anche nell'epoca dell'i.Pod.

corale della mozione n. 1-00031 presentata da me come prima firmataria sulla cultura, la formazione e i libri, che invita il Governo ad adottare misure finalizzate al recupero delle risorse per avviare campagne per la promozione della lettura, anche attraverso incentivi fiscali all'acquisto del libro, coinvolgendo famiglie, scuole e società in progetti che incoraggino i giovani a questa pratica, che le statistiche ci dicono, anno dopo anno, sempre più in calo, anche se in termini percentuali disomogenei nei diversi Paesi dell'Unione europea. ad assumere iniziative che agevolino la circolazione di idee e dei contenuti culturali che il nostro Paese va progressivamente elaborando; a prevedere un sostegno agli investimenti tecnologici su tutta la filiera commerciale (editori, distributori, grossisti, librai) per favorire l'adozione di strumenti moderni di gestione; ad arginare la deriva culturale, la superficialità, l'effetto trainante della massificazione (soprattutto grazie a certi spettacoli) che dilaga fra le giovani generazioni e che è in assoluta controtendenza con la storia del nostro Paese che il mondo intero ci invidia. Infine, ed è l'elemento a cui faccio riferimento in maniera più puntuale, impegna il Governo a verificare la possibilità di rendere la spesa per i libri di testo scolastici

veniamo sempre mortificati da tutte le parti: dal Presidente di turno, dalla stampa che tutti i giorni comincia la solita solfa che non facciamo niente. essere tutti solidali, *in primis* i Presidenti, nel difendere l'operato dei parlamentari che ci stanno e che lavorano. È ora di finirla anche con certi giornali della sinistra dei miei stivali che la fanno sempre lunga con le questioni dell'inattività e dell'improduttività dei parlamentari. Signora Presidente, mi rivolgo a lei, perché non ne posso veramente più. Qui manca qualcosa che probabilmente tutti quanti conosciamo molto bene: manca l'organizzazione dei lavori e manca la produttività. Ma non è certo colpa nostra se non c'è la produttività, perché il lavoro c'è, e non viene fatto solo in quest'Aula, ma anche a casa, sul territorio e dovunque, dai parlamentari seri che lo fanno seriamente. È ora di finirla, quindi.

Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, il provvedimento in esame individua un punto di equilibrio tra le posizioni e gli interessi dei diversi operatori della filiera del libro (editori e librai, grandi e piccoli) tutela inoltre gli interessi dei consumatori, garantendo l'accesso all'acquisto di libri a prezzi corretti. Attualmente il settore del libro è in forte crisi. La garanzia di condizioni che favoriscano una platea più vasta di librai ed editori contribuisce allo sviluppo del settore librario, tutelando al contempo il pluralismo dell'informazione. Il disegno di legge in esame attribuisce all'editore e all'importatore il diritto di stabilire il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale e limita al 15 per cento lo sconto praticabile sul prezzo di vendita, indipendentemente dalle modalità di vendita. L'editore e l'importatore potranno realizzare campagne promozionali che, per un periodo non superiore a un mese, prevedano sconti a vantaggio del consumatore finale, fatta salva la facoltà del rivenditore al dettaglio di non aderire a tali campagne. Può essere praticato uno sconto massimo del 20 per cento. Si escludono dalla disciplina in materia di prezzo di vendita al dettaglio e di sconti alcune categorie particolari di prodotti librari, quali libri per bibliofili, libri d'arte, libri antichi o edizioni esaurite, libri usati, fuori catalogo, pubblicati da almeno 20 mesi, edizioni destinate a rapporti associativi o libri venduti attraverso il commercio elettronico. Si prevede l'ipotesi di prezzo complessivo di collane, collezioni o grandi opere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi, mentre si esclude l'applicazione di norme in materia di vendite promozionali alle vendite di libri. La legge aiuterà il settore dell'editoria, attraverso l'adozione di un modello europeo intermedio, simile a quello francese. La regolamentazione delle campagne promozionali è un altro aspetto importante. Tra un anno sollecitiamo il Governo a procedere a una verifica sullo stato di applicazione della norma. C'è un vasto consenso nei confronti di questa iniziativa legislativa, ma il mondo delle librerie, dei librai e delle case editrici è estremamente variegato con realtà regionali particolari e situazioni diversificate, che necessitano di monitoraggio. importante dunque che le intese raggiunte sul tema dello sconto siano monitorate con attenzione anche dall'Autorità *antitrust*. La promozione del libro rappresenta uno stimolo positivo per la cultura in generale. Annuncio, quindi, il voto favorevole al provvedimento da parte della Lega Nord.

che si è creato attorno a questo progetto di legge, non credo siano necessarie molte altre parole per illustrarne i contenuti e i positivi riflessi che ci aspettiamo che esso produca nel vasto e complesso mondo del libro. Esclusa la scelta di parlare del merito di questo progetto di legge, mi soffermerò, dunque, signora Presidente, sul metodo con il quale esso è stato preparato, elaborato, discusso emendato sino a giungere, nella sua forma finale, a questo nostro voto di oggi nell'Aula del Senato. È questo un progetto di legge che viene da lontano. Non solo e non tanto perché esso si innesta su una previsione di legge di dieci anni fa (articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62), ma perché, nella forma che è oggi sottoposta al nostro voto, esso è il frutto di uno sforzo durato quasi cinque anni. Il punto di partenza di questo lavoro va, infatti, ricercato nel lavoro teso a produrre un'organica riforma del settore dell'editoria avviato dal Governo Prodi per impulso, e sotto la responsabilità dell'allora sottosegretario

All'interno di quella complessiva riforma, che giunse sino all'approvazione da parte del Consiglio dei ministri e che, come disegno di legge, venne successivamente presentato alla Camera per poi decadere insieme alla legislatura, un capitolo specifico era per l'appunto destinato a regolare il meccanismo di formazione del prezzo del libro, come ormai sappiamo un elemento centrale nel definire la natura stessa dell'intera filiera del libro. Alla scrittura della parte destinata, per l'appunto, a regolare il sistema di formazione del prezzo del libro, si era arrivati, così come per il resto del disegno di legge di riforma dell'editoria, dopo e attraverso una lunga, dettagliata e vasta consultazione che, prima su Internet e poi attraverso una corposa serie di audizioni, aveva coinvolto tutte le componenti del mondo del libro e, da ultimo ma certo non per ultimo, aveva visto un protratto e positivo confronto con le competenti Commissioni parlamentari. Con la nuova legislatura, enucleata dal resto del provvedimento originariamente destinato a riformare il mercato editoriale, la parte specificamente concentrata sul prezzo del libro è stata ripresentata come autonomo progetto di legge dallo stesso onorevole Levi, che ne è stato il primo firmatario e che su di esso ha raccolto la firma di molti colleghi di diversi Gruppi politici. Su questo testo, presso la Commissione cultura della Camera e in un dialogo stretto con le associazioni rappresentative del settore del libro, prime tra tutte l'Associazione italiana degli editori (AIE) e l'Associazione dei librai italiani si è sviluppato un intenso dibattito che, con il coinvolgimento e l'ascolto delle autorità indipendenti di controllo competenti in materia, della direzione generale per la concorrenza della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha, infine, portato all'adozione all'unanimità in sede legislativa del testo che è stato poi trasmesso a noi senatori. A questo punto, per quanto vaste e pubbliche fossero state le consultazioni e il dibattito, si è sviluppata - a nostro avviso positivamente una ulteriore e vivace discussione che ha visto tra i più attivi protagonisti parti del mondo del libro, librai ed editori minori, che non si sono pienamente riconosciuti nel testo prodotto da quelle consultazioni e da quel dibattito. Operando largamente con i più nuovi strumenti della comunicazione elettronica, questi soggetti sono efficacemente riusciti a far sentire le loro voci e le loro ragioni tanto all'interno del mondo del libro quanto all'interno del Parlamento. Si è così aperta una nuova fase di discussione che, di nuovo, col coinvolgimento di tutte le componenti del mondo del libro e in stretta collaborazione tra le Commissioni pubblica istruzione e cultura di Senato e Camera e sotto la guida dei rispettivi Presidenti - e qui voglio ringraziare il presidente Possa ha finalmente portato, dopo un decisivo confronto con il Governo, alla condivisa elaborazione del testo oggi sottoposto al nostro voto. Mi sento, dunque, in conclusione di dire che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che, se non per i suoi tempi, certo per il merito e per il metodo, costituisce un esempio di buona legislazione, di dialogo proficuo tra le forze in Parlamento. Un particolare ringraziamento va anche ai colleghi Vita e Asciutti per il lavoro svolto. La difesa delle piccole e medie librerie, delle case editrici di minori dimensioni, che questo disegno di legge si propone, in un Paese - l'Italia - che condivide con la Grecia il triste primato di più basso livello di consumi culturali, è un obiettivo importante. Credo, insomma, che votando ed approvando oggi, come mi auguro e confido, tutti insieme questo disegno di legge, si possa serenamente dire che la politica questa volta ha fatto bene la sua parte e ha scritto una pagina positiva.

in qualche modo incrinare questa comunione di intenti, ma lo faccio perché credo vada consegnata alla storia della Repubblica italiana la resistenza di un minimo di approccio liberale e liberista nei confronti della sacra e santa unione tra editori, librai e le maggiori organizzazioni di rappresentazione degli utenti e dei consumatori, che non necessariamente sono passate alla storia per fare gli interessi degli stessi.

in un luogo dove il dibattito si faccia a e 360 gradi, sulla base della lettura tanto sbandierata all'interno di questo documento. Visto che si parla di lettura, che si è parlato di pluralismo culturale,

«Per promuovere la lettura, come leva per l'innovazione e lo sviluppo economico e sociale del Paese, dove i dati sopra indicati evidenziano un livello molto basso di «lettori», il presente disegno di legge s'inserisce in un quadro dove la cultura e la protezione dell'editoria - veicolo di fruizione del sapere - devono prevalere, invece, sulle pure logiche del mercato. Fissare il prezzo dei libri significa allora - almeno per un po' - gestire il forsennato capitalismo liberista...».

«per salvaguardare la cultura nella sua forma più ampia». Io credo, proprio perché ritengo che la cultura più ampia includa anche il liberalismo, che occorra astenersi su questo disegno di legge. «Perché il prezzo assume un ruolo persino superiore al suo oggetto, quasi una metafora del tema dei saperi: del resto, il diavolo s'incarna nei particolari». Spero, quindi, che alla Camera decidano con buon senso di aprire un dibattito su questa tematica. Ricordo a tutti coloro i quali sono a favore o contrari al «forsennato capitalismo liberista» che solo là dove esiste la libertà garantita anche dalla legge esiste la possibilità di scambiare le idee e di far arrivare a conoscenza anche quelle della nicchia più piccola. Tutto il resto, se posso anch'io fare un po' di controcultura a buon mercato e un tanto all'etto, è Enciclopedia sovietica.

*relatore*. Signora Presidente, signori del Governo, colleghi, il disegno di legge n. 2146, d'iniziativa della Lega Nord, arriva in seconda lettura, essendo stato approvato in sede legislativa dall'altro ramo del Parlamento. Esso riguarda la Biblioteca italiana per ciechi di Monza, un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale che persegue lo scopo di avvicinare alla lettura le persone minorate della vista. La Biblioteca sostiene, attraverso servizi di trascrizione e di consulenza, l'integrazione di circa 3.000 studenti non vedenti delle scuole di ogni ordine e grado. Tra le finalità della biblioteca c'è anche un'attività informativa e divulgativa. Il patrimonio librario in linguaggio Braille destinato alla lettura vanta oltre 6.000 opere di autori italiani e stranieri, nonché un'ingente produzione su supporto informatico. L'istituto è anche impegnato fortemente nella trascrizione in linguaggio Braille di opere e di spartiti musicali, e ha ricevuto per tale attività importanti riconoscimenti internazionali. Il principio al quale si ispira la Biblioteca è quello di fornire libri scolastici effettivamente accessibili e fruibili, adattando e personalizzando quelli in uso nella scuola e nelle facoltà universitarie. Il disegno di legge, originariamente presentato alla Camera, prevedeva l'assegnazione di un contributo pari a 7 milioni di euro a decorrere dal 2009. Il testo al nostro esame, invece, prevede all'articolo 1 che il contributo, fissato dalla legge n. 260 del 2002 in 4 milioni di euro, sia incrementato di un importo pari a 600.000 euro per il 2010, a 700.000 per il 2011 e infine, a 1.682, 90 euro a decorrere dal 2012.

L'articolo 2 del disegno di legge interviene sull'articolo 3 della legge n. 52 del 1994 con riferimento alle attività della Biblioteca. L'articolo 3 invece si occupa della copertura finanziaria. 7a Commissione ha iniziato l'esame il 7 luglio scorso. Il 15 settembre si è concluso il dibattito. Le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso parere non ostativo sul testo nelle sedute del 28 settembre e del 6 ottobre 2010. In particolare, nella seduta del 5 ottobre la Commissione bilancio rilevava la necessità che il Governo confermasse la sussistenza delle risorse, tenuto conto che la certezza degli stanziamenti risaliva all'aprile 2010. Il 6 ottobre, il sottosegretario Casero ha confermato l'esistenza della dotazione economica a copertura del provvedimento. Il 23 novembre 2010, la 7a Commissione ha concluso l'esame in sede referente col voto favorevole di tutti Gruppi, registrando peraltro la piena disponibilità dei diversi schieramenti a richiedere il trasferimento in sede deliberante. Il 2 dicembre è stata avanzata formalmente la richiesta alla Presidenza del Senato. Il Governo ha comunicato il diniego a tale trasferimento poiché, secondo la Ragioneria generale dello Stato, l'autorizzazione di spesa prevista dal provvedimento per la copertura degli oneri è stata definanziata ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. L'*iter* del provvedimento si è così bloccato in attesa di una nuova copertura.

Oggi, su «L'Osservatore Romano» è riportata questa citazione, mentre si ricorda che è possibile per i ciechi e i sordi visitare la Biblioteca e i Musei vaticani. Credo che ciò sia in sintonia con quanto stiamo facendo oggi. Anche noi, quindi, siamo chiamati a contribuire in maniera concreta e significativa

- ha cercato di soddisfare le esigenze culturali e di apprendimento degli ipovedenti e dei non vedenti, oltre ad essere

a potenziare, anche dal punto di vista economico, l'altissima professionalità delle persone che lavorano all'interno di questa Biblioteca. Possiamo dire che «si può dare di più» ed abbiamo scelto di farlo: incrementare le risorse a sostegno della biblioteca significa offrire maggiori opportunità. Per dimostrare l'enorme impatto sociale che deriva dall'assegnazione di maggiori contributi, ma soprattutto per dare la percezione tangibile della realtà delle persone

il dato riportato dal Ministero della salute - quindi, un dato per noi oggettivo - parla di un aumento del 30 per cento di ipovedenti e non vedenti negli ultimi 20 anni,

molto bello poter dare oggi una risposta anche alle istanze di questa mamma, che scrive: «Gentile ministro Bondi, mi rivolgo a lei per fare un appello in favore della Biblioteca italiana per ciechi e ipovedenti "Regina Margherita" di Monza, affinché non vengano applicati i tagli previsti dallo Stato sui fondi destinati annualmente ad essa. Sono la mamma di un bambino ipovedente di 11 anni. Essere ipovedente significa vedere meno di tre decimi e che questa minorazione visiva non è correggibile in nessun modo. L'ipovedente ha un percorso di vita per certi aspetti ancora più difficile rispetto ad un cieco. Il cieco, infatti, si vede che è cieco, e questo, nella maggior parte dei casi, è sufficiente a garantirgli il rispetto e la comprensione degli altri. Per l'ipovedente invece non è cosi. Spesso passa per un maleducato perché non saluta, quando semplicemente non riesce a vedere bene le fattezze della persona che gli passa accanto. A scuola sembra distratto - e pertanto rimproverato - solo perché il suo sguardo sembra vagare nel nulla. Tra le tante difficoltà che un ipovedente deve affrontare c'è quella del diritto allo studio. Ora che è alla scuola media, e che non è più possibile dotarlo dì testi cartacei ingranditi,

che tengano in considerazione queste variabili personali dovute alla disabilità visiva. La Biblioteca di Monza, peraltro, oltre ai testi scolastici vanta una discreto numero di libri di narrativa e saggistica in formato Braille e a caratteri ingranditi, i quali permettono ai ciechi e agli ipovedenti di avere accesso alla cultura più in generale. Lo ribadisco, senza questi ausili, senza il necessario servizio che offre la Biblioteca di Monza, molti ciechi e ipovedenti si vedrebbero negati

mamma vede trovare una risposta, oltretutto all'unanimità, alla sua richiesta. Non so a voi, ma a me, quando l'ho letta, ha fatto venire «la pelle d'oca» pensare che una mamma debba rivolgersi ad un Ministro per vedere vedere riconosciuto il diritto allo studio. Ogni mamma spera che il proprio figlio studi e raggiunga obiettivi grandiosi e importanti per la sua vita. Credo quindi che quello che oggi oggi facciamo abbia un valore sociale e culturale: il nostro obiettivo e la nostra aspirazione deve essere quella di creare le condizioni affinché anche un ipovedente o un cieco possano vivere quelle emozioni emozioni subliminali che noi normodotati abbiamo la possibilità dì provare di fronte, ad esempio, al «Giudizio universale» di Michelangelo, o leggendo un grande romanzo come i «Promessi Sposi», oppure continuando a leggere e rileggere l'opera di Dante. È una questione di uguaglianza. È il segno di un Paese civile come è e vuole essere l'Italia. In seconda battuta, tutto ciò si traduce nella creazione diretta di prospettive di lavoro. La cultura, la formazione scolastica e quella universitaria possono consentire agli ipovedenti e ai non vedenti di accedere al mercato del lavoro, di realizzarsi anche sotto questo profilo e di non essere assistiti dallo Stato. La loro dignità ci chiede questo. Lo Stato non deve quindi limitarsi a fornire solo una assistenza materiale, indispensabile ma non sufficiente.

«Secondo me non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo, ciechi che vedono, ciechi che, pur vedendo, non vedono!» Noi oggi - oltre a rispondere alla mamma

Signora Presidente, colleghi, condividendo i contenuti già espressi dal relatore, vorrei cogliere l'occasione per sottolineare anch'io l'importanza dell'opera svolta dalla Biblioteca «Regina Margherita» di Monza, come anche da altri istituti e associazioni che su tutto il territorio italiano si impegnano per migliorare la qualità della vita di ciechi e ipovedenti. Promuovere la cultura e la conoscenza e far sì che anche i diversamente abili possano usufruirne è un dovere che il legislatore Costituente ha inteso inserire nella nostra Carta fondamentale. Questa attività di promozione è svolta da tempo dalla Biblioteca per ciechi «Regina Margherita» di Monza, che persegue lo scopo di avvicinare alla lettura - rendendo fruibili i normali testi cartacei - le persone minorate della vista. Numerosi studenti con problemi gravi alla vista sono infatti messi in condizione di apprendere, grazie all'opera di trascrizione e digitalizzazione delle opere da parte della Biblioteca. La Biblioteca ha un patrimonio letterario importante, con migliaia di opere all'attivo. Essa garantisce la fruibilità di testi per le scuole di ogni ordine e grado, università incluse. Infatti, in virtù di accordi con gli editori, la Biblioteca riceve il formato digitale dei testi da loro editi e si adopera al fine della indicizzazione, della trascrizione in testo ingrandito e della conversione del testo in Braille. Infine, ma non certo in ordine di importanza, la Biblioteca favorisce lo sbocco occupazionale per i minorati della vista, proprio tramite la suddetta opera meritoria di trascrizione dei testi in linguaggi utili. Da qualche tempo a questa parte, detto lavoro di trascrizione si è rivolto anche verso opere e spartiti musicali, non senza conseguire importanti riconoscimenti internazionali per l'opera svolta. Anche in ragione dell'aumento significativo della richiesta di testi su supporto cartaceo o digitale e in conseguenza della mole di lavoro che l'istituto si si trova a svolgere o, in alcuni casi, nell'impossibilità di svolgere, oggi - immagino all'unanimità - rivedremo la legislazione relativa al contributo in favore della Biblioteca «Regina Margherita». Le norme intervenute sino ad oggi sono state numerose ma, come detto, abbisognano di una rivisitazione. Al di là dello stanziamento economico in favore dell'istituto, all'articolo 2 si disciplina la possibilità da parte dell'istituto di stipulare apposite convenzioni con biblioteche e centri di produzione, per assicurare un servizio più adeguato. facoltà già esistente nel nostro ordinamento, alla quale si associa quella di potenziare la rete dei centri di consulenza tiflodidattica, allo scopo di garantire la copertura dell'intero territorio nazionale. un fine davvero molto importante perché, come meglio dirà il collega Giambrone, ci risulta che, in seguito ad atti amministrativi del Ministero dell'istruzione, istituti scolastici con le stesse caratteristiche e finalità della biblioteca in questione, non siano più in grado di garantire le nuove iscrizioni per l'anno scolastico 2011-2012. Per tutti questi motivi - e mi avvio a concludere, signora Presidente - mi auguro che il provvedimento in questione possa essere licenziato oggi stesso da quest'Assemblea e che lo stesso possa trovare attuazione nel più breve tempo possibile. Auspico anche che, vista la sensibilità del Parlamento verso l'argomento, si possa aprire una riflessione e trovare un modo per riconoscere e finanziare anche le tante associazioni ONLUS e di volontariato che, in maniera capillare in tutta Italia, svolgono compiti, servizi e funzioni di grande utilità sociale a beneficio delle persone con disabilità. *(Applausi

Questo è il dato più importante e significativo. Per primi, alla Biblioteca italiana «Regina Margherita» di Monza, ci si è posti il problema della pubblicazione di libri la situazione quando si doveva comporre un libro o un volume usando la semplice tavoletta e il punzonatore: si poteva fare un libro alla volta, con molta lentezza. La Biblioteca «Regina Margherita» ha invece sempre seguito l'evolversi delle varie tecnologie e delle varie tecniche; siamo passati quindi dall'edizione del volume singolo, via via negli anni, con tecniche e tecnologie sempre più sofisticate, ad una produzione di volumi su larga scala. Poiché tutti noi, quando pensiamo alla biblioteca, pensiamo ad un luogo dove si conservano i libri, io vorrei invece rilevare come questa sia stata una biblioteca che si è preoccupata della diffusione dei libri ad un particolare gruppo di cittadini. Se a noi sfuggisse questo elemento, dovremmo chiederci perché finanziare una biblioteca che in fondo ha sede in una città, come ce ne sono altre. Invece, non ce ne sono altre di biblioteche così; non ci sono altre biblioteche che hanno svolto l'attività della Biblioteca «Regina Margherita» di Monza. Ricordo che, fin dagli inizi, altre istituzioni che sono nate in città pur prestigiose per quanto riguarda la cultura - ricordo che la prima biblioteca «Regina Margherita» è nata a Firenze - non

la loro capacità di dare risposta ai problemi della gente. Questa sera noi siamo qui ad occuparci di una istituzione che ha un rilievo di carattere nazionale. Certo, essa risponde a molti problemi di cittadini sul territorio monzese e sul territorio milanese: ma questa non è l'unica attività che svolge. Non solo: oggi la Biblioteca, che è in grado di produrre su tutti i più moderni supporti e con tutti i più moderni sistemi (dall'edizione in Braille ai supporti audiologici), si sta anche

con l'evolversi della tecnologia, il Braille ha un futuro? È destinato ad essere ancora rilevante nella formazione dei ciechi?

che, alla luce delle moderne tecnologie, il Braille è destinato ad una involuzione e ad una chiusura lenta della propria storia, e chi invece sostiene che il Braille è ancora fondamentale per acquisire strumenti autonomi di cultura da parte dei ciechi, soprattutto da parte dei giovani che si accostano agli studi e al mondo della cultura. della cultura. In questo Paese spesso si insiste molto su quanto la scuola italiana abbia favorito il processo di integrazione degli allievi portatori di qualche disabilità. Questo è un settore dove ciò è molto difficile. È vero ‑ come diceva la collega che mi ha preceduto un ragazzo cieco; ma, in realtà, il ragazzo cieco è portatore di una disabilità che a volta mette a disagio la scuola, perché egli non ha una disabilità intellettiva, non ha una disabilità culturale e non ha una disabilità motoria. Ha una disabilità che è in grado di inquietare e di porre domande cui spesso i docenti non sanno rispondere. Ricordo in anni lontani, quando ancora insegnavo al liceo classico, di aver avuto uno studente cieco. Sapete cosa vuol dire per uno studente cieco fare una traduzione dal greco utilizzando quel mitico vocabolario che è il «Lorenzo Rocci»

noi parliamo spesso di integrazione, ma non ci rendiamo conto dei grandi problemi che l'integrazione porta dentro la scuola italiana: problemi che devono essere risolti. Anche su questo punto, la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza ha dato un contributo significativo, perché è all'avanguardia per quanto riguarda i supporti didattici, e perché è all'avanguardia anche per le forme di consulenza agli insegnanti e alle scuole e per l'inserimento dei ciechi dentro la scuola italiana. Questa Biblioteca, un organismo statico. Non è solo il luogo della conservazione del sapere; non è solo il luogo della conservazione dei libri. È una istituzione molto dinamica dal punto di vista del sostegno alla didattica, la Biblioteca ha fatto molto. Infine, ricordo un altro aspetto molto importante. Sono diversi, i soggetti diversi, i soggetti ai quali la Biblioteca si rivolge: i ciechi, i docenti della scuola, ma anche gli adulti che hanno a che fare con il mondo dei ciechi e degli ipovedenti, i genitori tutti quelli che si occupano di questi argomenti. Anche a loro la Biblioteca ha riservato una attenzione particolare, ed ecco perché si tratta di un'istituzione molto dinamica sul territorio, che

quanto può portare sempre più lontano nel sostegno e nella risposta ai bisogni, non solo solo di un gruppo di cittadini che, purtroppo, ha il difetto fisico di non poter vedere, ma anche di tutti gli altri cittadini che intorno a questo gruppo ruota e che, con i propri figli, i propri studenti, i propri amici, vuole dare risposte sempre più compiute e sempre più importanti per l'inserimento sociale, per l'inserimento culturale

su come tutti questi servizi, così importanti dal punto di vista sociale - ma così importanti dal punto di vista nobile del termine solo in alcune aree del Paese. Questo è un problema: è come se, nel Paese, a volte vi fosse difficoltà ad avere, in aree

perché questo tipo di servizi, anche di elevato valore tecnologico e scientifico, siano fruibili da

offrire a tutti i cittadini gli stessi servizi e, se possibile, un livello accettabile di qualità di questi servizi. Noi siamo qui oggi ad esaminare una realtà;

che i cittadini hanno di tutte queste istituzioni così importanti. Questo, infatti, è un caso in cui la distanza geografica può fare ancora molto la differenza. Credo che

intervenute. Dal tono dei loro interventi si evince una condivisione di massima sul provvedimento: quindi auspico una votazione rapida e condivisa sul testo.

siano finanziate associazioni ONLUS che si occupano di persone con disabilità. È un auspicio che facciamo tutti. Mi auguro che quanto prima si riescano a trovare i finanziamenti per poterlo fare. infine la senatrice Mazzuconi che ci ha voluto ricordare che si tratta di una biblioteca di assoluto rilievo nazionale, anche se ha sede soltanto a Monza. La

nel merito si condivide senz'altro la finalità di fondo perseguita dal provvedimento in esame, che intende potenziare l'attività di questa biblioteca, che svolge una meritoria attività di sostegno alle persone non vedenti e ipovedenti, nonché un'attività di organizzazione dei servizi diretti

di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222"; che all'articolo 3 comma 1, le parole: "bilancio triennale 2010-2012" siano sostituite dalle altre: "bilancio triennale 2011-2013"; - che all'articolo 3, comma 1 le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010" siano sostituite dalle altre: "Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011"».

Il provvedimento in questione è stato già approvato, peraltro in sede deliberante, dai parte dei colleghi della Camera dei deputati. La Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, persegue da tempo lo scopo di avvicinare alla lettura le persone minorate della vista, garantendo loro un importante strumento di svago e di crescita culturale. Detta biblioteca garantisce appunto - grazie ai suoi servizi - l'integrazione dei circa 3.000 studenti non vedenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre che svolgere un'attività informativa e divulgativa. Come già evidenziato dai colleghi in sede di discussione generale, la legislazione di riferimento è ampia:

Come già accennato e come descritto da numerosi colleghi prima di me, l'opera svolta da questa biblioteca è vasta oltre che meritoria. Essendo aumentata negli ultimi anni la domanda di testi su supporto cartaceo o digitale, l'impegno della biblioteca si è accresciuto notevolmente. Più di 3.000 libri vengono trascritti, digitalizzati, resi fruibili ogni anno scolastico. La biblioteca si preoccupa, infatti, di rendere fruibili i testi cartacei in uso nelle scuole e nelle università. L'istituto, in virtù di un accordo con gli editori, acquisisce le copie digitali dei libri assumendosi per intero l'onere di rielaborarlo, in applicazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, mediante modifiche atte a consentire la stampa in linguaggio Braille o in caratteri ingranditi ovvero per consentirne la lettura con il sintetizzatore vocale. La biblioteca contribuisce in modo rilevante alla formazione ed alla ricerca di sbocchi occupazionali per i non vedenti. Annunciamo il nostro voto convinto a favore del provvedimento in questione, cercando l'attenzione dei colleghi senatori e del Governo su altri istituti scolastici in cui, a seguito dei famosi tagli lineari, signor Sottosegretario, dell'attuale Esecutivo, questa opera di promozione e divulgazione del sapere, per i soggetti diversamente abili a causa di *deficit* della vista, non potrà più avvenire a partire dal prossimo anno scolastico. Ho provveduto alla presentazione di un atto di sindacato ispettivo al riguardo, sul quale spero ci sia da parte del Ministro, oltre che la volontà di rispondere celermente (questo quanto meno per garantire agli utenti la conoscenza del problema), la promessa di trovare una soluzione pratica ed in tempi utili al fine di permettere ad altri istituti - così come dicevo - presenti sul territorio italiano di continuare ad accettare le iscrizioni per il prossimo anno scolastico,

intende potenziare l'attività della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza, la quale rappresenta uno dei centri di eccellenza nel settore dei servizi culturali ai non vedenti. Permettetemi altresì di evidenziare l'esigenza di adeguare i servizi di pubblica lettura alle necessità dei gruppi minoritari, tra i quali quelli rappresentati dalle persone con disabilità sensitivo-motorie che non possono usufruire dei servizi principali. Si rende pertanto necessario adottare ulteriori

l'attività del Centro Internazionale del Libro Parlato di Feltre, istituito nel 1983, con lo scopo di aiutare i non vedenti ad accostarsi alla lettura ed allo studio. Al Centro si rivolgono esclusivamente non vedenti, ipovedenti, dislessici, distrofici, anziani, malati terminali e tutti coloro per i quali la lettura in modo tradizionale non è possibile; già la legge 3 agosto 1998, n. 282 ha stanziato un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, e al Centro Internazionale del Libro Parlato di Feltre; un altro centro nazionale specializzato nel settore è rappresentato dalla Biblioteca Italiana per ipovedenti «B.B.I. Onlus» di Treviso, che negli ultimi anni ha conseguito un esplicito riconoscimento dell'importanza culturale e sociale delle attività svolte in ambito regionale e nazionale; l'attività della Biblioteca italiana per ipovedenti «B.B.I. Onlus» di Treviso è sottoposta alla vigilanza del Ministero beni e attività culturali;

istituita alla fine dell'Ottocento, prima con sede a Firenze, poi a Genova, poi a Milano. Per ripararsi dai bombardamenti, arrivò infine a

di tutta evidenza che ci sono altri centri collegati in giro per l'Italia, e l'articolo 2, tra l'altro, prevede convenzioni con enti locali ed istituzioni affinché si possa dilatare a rete i servizi che tale biblioteca offre.

è il prodotto che rende le persone ipovedenti e cieche cittadini che hanno il diritto alla formazione e all'istruzione fino al massimo grado, come tutti gli altri cittadini italiani. è stato insegnante ha spiegato quanto sia difficile, nonostante i sussidi e i supporti, poter integrare effettivamente la persona che ha una menomazione visiva.

di poterlo avere sul comodino la sera prima di dormire. Senza il libro Braille moltissimi tra coloro che amano la cultura, a cui noi vogliamo offrire continuità di acculturazione, non avrebbero questo strumento tra le mani. Pertanto, oltre a tanti altri meriti, soprattutto quello di fornire testi scolastici, questa istituzione mette le persone, non vedenti o ipovedenti, nella condizione di di fruire dei frutti della civiltà letteraria ed artistica di questo Paese. Lo dobbiamo a loro, perché ne hanno diritto, ma lo dobbiamo anche alla tradizione culturale del Paese. Ecco perché, che ci sia un finanziamento nazionale e che ci sia un'ulteriore integrazione di un finanziamento che si era ridotto è una necessità. È doveroso farlo, ed è bello che in proposito ci sia un consenso unanime. *(Applausi dai Gruppi*

il Popolo della Libertà dichiara il pieno consenso a questa proposta di legge di iniziativa parlamentare, che aumenta il contributo dello Stato a favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, incrementandone altresì le tipologie di attività. Al riguardo, va apprezzato il Governo che, nelle attuali e ben note difficoltà di bilancio dello Stato, è riuscito a reperire in «zona Cesarini» - diremmo noi - le risorse necessarie per la copertura del provvedimento. Come ha ben sottolineato il relatore, senatore Bevilacqua, e come hanno efficacemente illustrato i colleghi intervenuti prima di me in discussione generale, la Biblioteca di Monza svolge da molti anni nel nostro Paese un'importante attività in favore dei minorati della vista. Consentite anche a me in sede di di evidenziarne l'importanza sociale, riassumendone gli elementi caratteristici. L'azione della biblioteca si rivolge a diverse tipologie di utenti, non vedenti e ipovedenti, scolari, studenti, cittadini.

migliaia. L'azione della Biblioteca di Monza riguarda la produzione di testi di letteratura amena (narrativa e saggistica, eccetera), di cui la senatrice Garavaglia ha poco fa sottolineato l'importanza, di testi di approfondimento personale

di testi musicologici e spartiti musicali e di testi scolastici e di studio. È soprattutto verso quest'ultima produzione di testi scolastici e di studio che si è orientata l'attività di produzione della Biblioteca di Monza di questi ultimi anni. Per ciascuno di questi tipi di prodotti, la biblioteca è in grado di realizzare varie versioni: la versione cartacea in Braille ad uso dei non vedenti; la versione cartacea a caratteri ingranditi ad uso degli ipovedenti; la versione digitale per sintetizzatore vocale e/o per *display* Braille, perché ultimamente sono saltate fuori anche nuove utilizzazioni digitali.

sempre adattata alle specifiche esigue capacità visive dell'alunno, della realizzazione; per la produzione di testi digitali il rapido sviluppo della tecnologia di questi ultimi anni con l'implementazione di varie opzioni La biblioteca dispone di un proprio catalogo di opere complete già pronte frutto di un'attività di circa 80 anni

Oltre ad essere organizzata in «centro editoriale» specializzato (sussidiario e non alternativo all'editoria comune), la biblioteca, per svolgere meglio il supporto scolastico agli alunni minorati della vista, si è strutturata territorialmente

una consulenza tiflodidattica, la biblioteca svolge su tutto il territorio nazionale. diffusa assicura la copertura del 90 per cento del fabbisogno nazionale di consulenza. Tali strutture territoriali offrono alla scuola il necessario supporto nell'individuazione dei singoli specifici bisogni dell'alunno ipovedente o non vedente e nella scelta dell'approccio didattico migliore in relazione alle capacità e potenzialità Complessivamente, il numero di addetti al servizio di trascrizione della biblioteca è stimato in 180-200 unità lavorative, in gran parte personale di elevata professionalità e conoscenze specialistiche in campo informatico, tiflologico e didattico. La biblioteca svolge attività per un numero di alunni non vedenti e ipovedenti nelle scuole di ogni ordine e grado, dagli asili nido alle università, numero totale di poco meno di 3.000 studenti ogni anno. Le richieste annuali sono di oltre 600 trascrizioni in Braille di testi scolastici,

Può essere interessante segnalare che il costo di trascrizione dei testi scolastici necessari in un anno per singolo alunno può arrivare, nel caso di trascrizioni in Braille, fino a quasi 30.000 euro, nel caso di trascrizioni a caratteri ingranditi per ipovedenti fino a oltre 10.000 euro e, infine, nel caso di trascrizioni in digitale, fino ad oltre 5.000 euro. Questa è l'importanza dell'azione di supporto che viene effettuata per questi nostri fratelli più sfortunati. Anche solo questi dati di estrema sintesi evidenziano l'importanza dell'azione sociale svolta dalla Biblioteca di Monza, in particolare a supporto degli scolari e degli studenti minorati di vista, e motivano il convinto voto a favore

Signora Presidente, non parteciperò al voto, e non perché, da radicale, non mi interessi dell'accesso a qualsiasi tipo di cultura per chi è disabile. In quanto iscritto e dirigente dell'associazione «Luca Coscioni», devo dire che da sempre ci battiamo perché anche i muti possano parlare, oltre che affinché i ciechi possano leggere. Sarebbe stata una felice coincidenza se questo disegno di legge fosse stato un emendamento al disegno di legge poc'anzi approvato, in cui si imponeva, con tutti i favori che sono stati fatti agli editori, la produzione

I numeri che ci avete sciorinato parlano al massimo - se la memoria non mi tradisce - di 10.000 volumi all'anno: per 10.000 volumi l'anno, 700.000 euro annui vanno a questa benemerita associazione, cui meriti sono stati individuati dal 1929 a non si sa quando, perché tutto è stato presentato con il tempo al passato.

alcuni di loro vogliono continuare a chiamarsi così). Uno di loro è un mio compagno radicale scomparso poche settimane fa: si chiamava Paolino Pietrosanti, e grazie a un incarico dell'allora ministro Rutelli nella scorsa legislatura stava proprio negoziando con gli editori l'imposizione della pubblicazione di una serie di testi anche con questi formati, quindi non esternalizzando cose inutili, perché il *file* di un libro da stampare a caratteri più grandi o da mettere su Internet non costa assolutamente nulla in più, né tantomeno trasferirlo a una macchina che lo stampi in Braille, a oltre cento anni dall'invenzione di questo codice. Questa è una medaglia al valore.

Signora Presidente, ringrazio il Sottosegretario che si è soffermato un momento, perché è di tutta evidenza che, oltre che a noi stessi, vorrei ricordare qualcosa al nostro Governo. Come è noto,

Sapeva di essere in pericolo e non aveva nemmeno la scorta. Questo dice anche la mitezza della persona e la volontà di testimoniare una scelta personale e nelle istituzioni a garanzia della libertà propria e di tutti. Nella mozione approvata qui, signor Sottosegretario, ricorderà che ci fu anche un comma aggiuntivo nel quale dicemmo: in questo quadro

ed è anche questo un passo verso il riconoscimento della testimonianza della maggioranza cristiana del Sud Sudan, che ancora adesso è vittima purtroppo di soprusi e - ahimé! - di situazioni precarie, al limite del terrorismo, contro i cristiani. il ricordo è commosso per chi ha già donato la sua vita per essere fedele a un'idea e a una fede. Ed è un ricordo per tutti noi, affinché gli impegni che ci assumiamo vengano poi opportunamente e tempestivamente onorati. *(Applausi Signora Presidente, desidero associarmi, anche a nome del Gruppo del Popolo della Libertà, alle parole della senatrice Garavaglia. Si tratta di un uomo che è un simbolo per la sua stessa vita, un uomo che rappresentava come Ministro delle minoranze religiose proprio la difficile situazione delle minoranze in quel Paese, e purtroppo non solo lì. Quest'uomo è stato ucciso. Io credo che

intanto per manifestare il nostro cordoglio per la morte del Ministro, ma anche e soprattutto per chiedere al Pakistan di rispettare realmente i

contro la cosiddetta blasfemia, che finisce per essere applicata in generale a coloro che non appartengono alla religione musulmana, o addirittura a coloro non consono a determinati canoni. Credo che sia molto importante su questo punto l'unità che ha manifestato il Senato già settimane fa e questa sera, e sono certo che il Governo saprà farsene interprete.

Stamattina l'aveva ricordato anche il ministro Maroni durante l'audizione che si è svolta alla Camera dei deputati. Credo che effettivamente la figura sia come come raramente capita di incontrarne, e una volta di più credo che quello che è successo sia l'esemplificazione di come la strada da percorrere sia quella della comprensione e di creare, per quanto possibile, un dialogo interreligioso. Di questo si sta occupando anche il Consiglio d'Europa, che a breve produrrà una mozione su questo tema. Io credo, come ha già detto il collega Malan, che il nostro Paese, attraverso il Governo, si debba impegnare a livello europeo per far passare determinati concetti. Questa'Assemblea si è già espressa. Ripeto però quello che deve passare è il concetto che ci deve essere un dialogo tra le religioni, che ci deve essere la libertà religiosa. Non deve passare il concetto che questo possa esistere attraverso attraverso la semplice accettazione di un multiculturalismo che spesso è sterile e non porta affatto ad una migliore convivenza tra le persone. una nuova finestra"). Onorevoli colleghi, la Presidenza si associa agli interventi della senatrice Garavaglia, del senatore Malan e della senatrice Boldi, in sintonia con quanto il Senato ha già più volte ribadito sull'importanza della libertà religiosa come diritto inviolabile dell'uomo.